poneva l'accento sull'inattendibilità dei dati formulati nel DPEF. Al riguardo occorre fare delle considerazioni di carattere generale.

in pericolo la tenuta del sistema, dei consumi e così via. Bisogna concentrare gli sforzi in questo autunno affinché tutte le risorse disponibili vengano impiegate non

dei limiti, perché un conto è uno scontrino, altro è evadere costantemente. Sull'evasione dell'IVA andrebbero fatti dei ragionamenti di carattere territoriale, perché se in Calabria si spendono 150 euro ogni 100 euro dichiarati e in Lombardia 105 ogni 100 euro dichiarati, è evidente che c'è un problema di evasione che arriva ai livelli della pandemia; è un dato che troviamo in diverse aree del Paese. Il tema va affrontato in maniera seria, e siamo tutti d'accordo; sappiamo che la prospettiva corretta è quella del federalismo fiscale. Nel frattempo sarebbe anche opportuno che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza organizzassero i controlli sulla base di tale dato, cioè della diffusione dell'evasione come fenomeno sul territorio. Se andiamo a vedere la tabella con i controlli, scopriamo che la maggior parte dei controlli vengono eseguiti in Lombardia, ossia nella Regione che, in percentuale, evade meno rispetto al resto del Paese. Sarebbe opportuno che anche nei controlli si facesse un po'

al nulla, perché noi abbiamo evidenziato le criticità, i dati oggettivi della nostra economia e della finanza pubblica e abbiamo formulato proposte precise, ma da parte della maggioranza e del Governo non c'è alcuna risposta e alcun contraddittorio. Ci si rifugia semplicemente dietro alla posizione espressa in questa sede dai rappresentanti del Governo e della maggioranza.

di un accrescimento delle esportazioni. Nulla dice, nulla propone e nulla decide per accrescere il livello dei redditi e i consumi, quindi la domanda interna. Noi riteniamo invece che andava fatto il contrario, e cioè che la nostra economia potrà riprendere il suo cammino e si potrà intercettare la ripresa se si sostengono i consumi, se si agisce sui redditi. Il presidente del Fondo monetario internazionale ha recentemente dichiarato che l'economia mondiale è in una situazione molto precaria, quindi non ha scommesso, come fa il Governo italiano, su una ripresa certa, che le politiche di sostegno, quelle adottate dai principali Paesi sviluppati, non vanno smantellate, altrimenti il rischio è di uccidere la ripresa. Lo stesso ministro Tremonti, ieri, ha parlato di previsioni incerte.

che hanno il carattere della precarietà, e solo su esse. Questo è il punto che contestiamo questo è il cuore del nostro giudizio critico. Sempre ieri, la presidente di Confindustria ha detto che la politica sarebbe distratta di fronte alla grave crisi economica

che abbiamo di fronte, bensì determini l'oggettivo aggravamento degli effetti sociali della crisi. È vero o non è vero, signor Presidente, signor Vice Ministro, che la disoccupazione nei prossimi mesi aumenterà vertiginosamente, di quasi due punti percentuali, rispetto all'attuale livello, che già ha registrato una crescita molto grave da alcuni mesi a questa parte? Si può licenziare una manovra di politica economica e di bilancio ignorando tale dato? Questo è uno dei quesiti che proponiamo. È vero o non è vero che la caduta del prodotto interno lordo, di 6-7 punti percentuali durante

e che esiste un problema di redistribuzione del reddito nel nostro Paese? È vero o non è vero che la pressione fiscale ha raggiunto un livello *record*

e perché dovrebbe dire che la politica economica che sta portando avanti non affronta questi problemi. Anche questo è un dato oggettivo, non è una mia opinione: non c'è una politica per affrontare i gravi problemi della disoccupazione, dei redditi e dei consumi, del controllo della spesa pubblica, cresciuta di tre punti percentuali nell'ultimo anno, e così via. Ma non ci siamo limitati a richiamare questi ed altri problemi, abbiamo formulato proposte precise. Non è vero, come qualcuno dice, che l'opposizione non ha una proposta; l'opposizione ha proposte che ha formulato con precisione in tutte le circostanze nelle quali si è discusso di politica economica, in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento. Non è vero, ad esempio, che in questo momento storico la riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali: questa riforma è necessaria e si può e si deve realizzare in questo momento storico. Non è vero che non si possa agire con la leva fiscale in senso redistributivo, affrontando il problema dell'eccessivo carico fiscale sulle famiglie, sui redditi da lavoro e da pensione. E potrei continuare. Ma, appunto, il Governo è fermo: basta leggere la proposta di risoluzione che proviene dalla maggioranza, che è volta a confermare quello che è stato detto a luglio, cioè niente. Questo è il punto: il Governo scommette su previsioni incerte, come ho detto, e sulle entrate derivanti dallo scudo fiscale e questo è tutto. Di fronte alla più grave crisi economica dal dopoguerra ad oggi,

delle finanze*. Signor Presidente, tenendo conto che già nell'intervento di ieri del Ministro dell'economia sono stati forniti dati e motivazioni che suffragano non solo la Nota di aggiornamento, ma anche la costruzione della finanziaria, poco ho da aggiungere rispetto a quanto già detto ieri più autorevolmente in questa sede. Tuttavia, prendendo spunto dalle ultime dichiarazioni del relatore di minoranza, senatore Legnini, qualche osservazione occorrerà pur farla.

il Governo non avrebbe assunto iniziative e che spenderebbe troppo poco per affrontare la crisi. Ma guardiamo che cosa è stato fatto negli altri Paesi del mondo, come la crisi è stata affrontata e se per caso il caso il contenimento della spesa pubblica in questa fase non sia un'azione virtuosa tale da rimettere in piedi il nostro Paese meglio di quanto accada altrove.

a salvaguardia dell'occupazione (mi riferisco principalmente alla massiccia dose - circa 8 miliardi in due anni - di risorse pubbliche destinate alla cassa integrazione).

cercano di togliere lo zampino quando c'è il rischio di sporcarsi le mani. Dunque, le risorse per gli ammortizzatori sociali ci sono. Quindi, il livello di spesa pubblica per il sostegno ai ceti più deboli è paragonabile a quello di altri Paesi. Certo, noi abbiamo evitato accuratamente di entrare con le mani nelle casse delle banche e di impossessarcene, come è stato fatto, per esempio, oltreoceano e in altri Paesi europei. Questo mi sembra assolutamente ovvio: da una parte, perché il sistema bancario deve essere un sistema di carattere privato e non pubblico; dall'altra, perché tutti ci ricordiamo i danni che nel nostro Paese derivavano da un sistema di banche controllate dall'operatore pubblico. Questo, a garanzia anche dello sviluppo futuro del Paese. la questione principale sollevata nelle osservazioni dell'opposizione è che da una parte è aumentata la spesa pubblica, dall'altra, però, si fa troppo poco. Come direbbe il poeta, «la contradizion che nol consente»: non si può dire, da una parte, che si spende poco e, dall'altra, che si spende troppo. Esaminiamo i due corni del dilemma. Si spende troppo: in realtà, la spesa pubblica è rimasta contenuta e sotto controllo. Certo, è cambiato il rapporto con il prodotto interno lordo, ma questo dipende dal fatto che esso è calato, e quindi il rapporto è cambiato. Ciò non significa che sia aumentata la spesa. D'altra parte, se la spesa fosse aumentata, perché ci sarebbero tante lamentele in ordine al contenimento della spesa in molti settori? Cosa, d'altronde, che abbiamo cercato di fare. Ed arrivo alla questione fondamentale: se vogliamo diminuire la pressione fiscale e quindi precostituire uno strumento per poter poi far procedere ad un tasso di sviluppo superiore possibile il Paese, è chiaro che non si scappa. Non si può pensare di diminuire le tasse "gratis": bisogna pensare di diminuire corrispondentemente la spesa. è la diminuzione della spesa, è chiaro che non ci si può lamentare quando si incontra qualche misura di tagli alla spesa. È singolare volere i due obiettivi contemporaneamente (più spese e meno tasse) e che poi, nel momento in cui vi è qualche, non riduzione di spesa, ma contenimento della dinamica espansiva della spesa, come nel caso del comparto degli enti locali o della spesa sanitaria, ci siano ampie proteste. In realtà, In realtà, se bisogna partecipare tutti all'azione di risanamento della finanza pubblica e della riduzione della spesa, non vi può essere un *free ride*, quello che in italiano si potrebbe tradurre "scrocco", verso questo tipo di soluzione, ma tutti in qualche modo devono parteciparvi. se aumentassimo la spesa pubblica o corrispondentemente diminuissimo le tasse o percorressimo entrambe le direzioni, ci troveremmo per lo meno in una difficoltà che è la seguente: aumentare l'indebitamento, con i rischi che sono noti a tutti, soprattutto in una fase nella quale l'indebitamento globale da parte di Paesi che poco accedevano al debito pubblico è cresciuto in modo esponenziale, quindi con difficoltà di copertura di questo indebitamento, oppure dovremmo prefigurare un tempo successivo nel quale aumenterà la pressione fiscale, quindi tutti gli operatori saprebbero che oggi magari hanno un vantaggio fiscale ma domani dovrebbero pagare molto di più, e pertanto sarebbero disincentivati dall'investire nel nostro Paese, cosa che noi vogliamo evitare nel modo più assoluto perché è chiaro che stiamo ancora sotto gli effetti della crisi, ma dobbiamo pensare al domani. E al domani come si pensa? Cercando di attrarre investimenti e di rendere il nostro Paese più attraente di quanto non fosse stato prima.

di strumenti automatici di incentivazione (che si sono dimostrati nel passato una sorta di idrovora, quindi in qualche modo vanno controllati), di rifinanziare gli strumenti di sostegno del reddito, di aumentare il potere di acquisto delle famiglie e cose di questo genere; cose sulle quali non si può non essere d'accordo, in linea di principio, salva la necessità di conciliare tali finalità con il quadro economico complessivo. Ripeto: non si può volere contemporaneamente la diminuzione della spesa pubblica, lo sviluppo del Paese, la diminuzione delle tasse e l'aumento della spesa: si tratta di obiettivi tra loro inconciliabili e difficili da realizzare da parte di qualsiasi Governo, Tutto ciò, ovviamente, unito (e questa è l'ultima parte della proposta di risoluzione) al richiamo ad una politica fiscale francamente vessatoria. ad esempio, alla tracciabilità dei pagamenti, al famoso registro clienti e fornitori, che in realtà era un sistema per recuperare reddito, ma non certo un sistema di amicizia tra fisco e contribuente, non certo un sistema che in qualche modo invogliava ad evitare l'evasione. Era un sistema che spingeva i contribuenti (e forse questo è stato uno degli effetti più deleteri del biennio precedente rispetto a quello del Governo attuale) ad espatriare e a mettere al riparo all'estero le proprie fortune, cosa che assolutamente, anche da un punto di vista etico, non credo sia assolutamente condivisibile. Quindi, occorre un rapporto con il fisco sicuramente più amichevole,

se l'opposizione fosse favorevole a trovare una linea di accordo per la definizione di reali misure di contenimento della spesa pubblica, il Governo non potrebbe che esserne molto contento.

scoppiettanti o pirotecnici, ma sono documenti che realisticamente, tenendo conto dell'andamento dell'economia, cercano di dare un segnale di stabilità al sistema economico e di finanza pubblica italiana. la scelta della prudenza e di rifuggire da un avventurismo che forse altri avrebbero applicato se fossero stati al Governo sia la linea che ci può portare a superare questa crisi e a nutrire una speranza di crescita negli anni futuri.

abbiamo ascoltato con attenzione, sia ieri che oggi, la relazione del ministro Tremonti, il dibattito che si è sviluppato e ciò che il Governo ha proposto in sede di Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria. La prima considerazione che ci permettiamo di fare è che non c'è nulla di nuovo sotto il sole e che la prudenza e il timore che hanno guidato e guidano l'azione del Governo sui temi di politica economica e finanziaria, da un lato, possono essere comprensibili perché il clima di incertezza determinato dalla crisi produce anche la necessità di osservare e conoscere meglio le dinamiche economiche nazionali ed internazionali per poter intervenire, dall'altro, però ci fanno anche comprendere

per adottare una serie di provvedimenti che vanno nel senso della riforma di alcuni elementi ormai incrostati dell'economia italiana. La Nota di aggiornamento presenta uno scenario economico leggermente migliore rispetto a quanto ci è stato detto a luglio con il Documento di programmazione il dato più evidente riguarda il miglioramento del prodotto interno lordo di 0,4 punti percentuali per il 2009 e di 0,2 punti percentuali nonostante quanto rilevi la Nota di aggiornamento, però, la Commissione UE ha previsto un peggioramento del PIL rispetto a maggio (meno 5 per cento rispetto a meno 4,4 ha previsto un miglioramento del PIL per la Germania e per la Francia, pur essendo Stati esteri che in senso assoluto hanno subìto la crisi in misura maggiore rispetto al nostro Paese; la differenza la fa la loro dotazione infrastrutturale, che ha consentito loro di far riprendere in maniera più veloce l'economia. La Nota evidenzia peraltro come il commercio, nel secondo semestre del 2009, abbia mostrato segnali di recupero, nonostante l'economia italiana punti molto Il drastico calo del commercio internazionale ha rappresentato per il nostro Paese un elemento oggettivamente preoccupante. Rispetto a questo, né la legge di sviluppo né la manovra estiva hanno prodotto, in un'ottica di sistema per il per il sostegno delle eccellenze italiane, misure in grado di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso l'esportazione di modelli imprenditoriali vincenti quali i distretti italiani. Molto si è detto sulla tutela dei prodotti *made in Italy*, ma di concreto poco si è fatto. La Nota sottolinea altresì come da gennaio ad agosto il prezzo medio del petrolio si sia attestato alla media di 55 dollari al barile. Le previsioni indicano un progressivo aumento nei prossimi mesi, il che determinerà un aumento anche dei prezzi dei prodotti alimentari. I prezzi delle materie prime e dei prodotti alimentari, dovuti al basso prezzo del petrolio per gli uni e alla bassa inflazione per gli altri, hanno attutito gli effetti negativi della crisi. Con la previsione di un aumento degli stessi, a rischio sono i consumi delle famiglie italiane. In tema di energia si potrebbero quindi subire sempre più le conseguenze negative di una politica energetica, quella italiana, per il momento orientata solo nelle intenzioni e non nei fatti alla diversificazione delle fonti energetiche. Si nota ancora molta confusione sulla reale volontà del Governo di reintrodurre nel nostro Paese l'energia nucleare. Le fonti rinnovabili, d'altronde, pur crescendo, non riuscirebbero mai a compensare la necessaria riduzione della dipendenza da fonti energetiche tradizionali come gas e petrolio. In questo scenario le intenzioni strategiche del Governo, negli ultimi mesi, sono state solo quelle di privilegiare un rapporto amichevole con la Russia per garantirsi la stabilità e la certezza delle forniture di gas, piuttosto che attuare politiche volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo delle fonti energetiche alternative. Il quadro macroeconomico proposto dalla Nota evidenzia inoltre come gli investimenti fissi lordi in macchinari ed attrezzature presentano un calo del 17,2 per cento nel 2009 (meno 16,5 per cento era previsto nel DPEF). La situazione dovrebbe migliorare (probabilmente grazie alla Tremonti-*ter*, che ha introdotto la detassazione degli investimenti in macchinari) nel 2010. La situazione del 2009 è però estremamente preoccupante, in quanto denota l'incapacità delle imprese di investire in nuova capacità produttiva, visto il calo della domanda da una parte e la carenza di liquidità dall'altra. La manovra d'estate ha introdotto una misura che prevede la deduzione dal reddito imponibile del 50 per cento della spesa sostenuta in macchinari ed apparecchiature. presentata con l'intento di essere uno strumento utile agli esercenti le attività commerciali (persone fisiche e società) presuppone che le imprese debbano conseguire un utile, sul quale poi verranno applicate le imposte. In pochi forse hanno tenuto conto del fatto che in un anno in cui presumibilmente molte delle attività commerciali subiranno gli effetti della crisi economica, saranno ben poche quelle che effettivamente conseguiranno un utile. La misura non ha peraltro l'attitudine ad affrontare un supporto concreto alle imprese: gli investimenti per un'impresa sono, sì, necessari; tuttavia, il principale problema che devono affrontare non è il fabbisogno di nuova capacità produttiva, ma il drastico calo della domanda. La misura quindi è inadeguata rispetto alla odierna collocazione nel mercato delle imprese, alla loro capacità di sviluppo e al calo di produttività dovuto al calo della domanda. Per quanto riguarda l'occupazione, la Relazione previsionale e programmatica corregge i dati del DPEF e sostanzialmente presenta un quadro meno peggiorativo in merito alla riduzione dell'occupazione. È comunque una situazione preoccupante e soprattutto non destinata a risolversi nel breve periodo. La sensazione è che questo dato sia destinato a salire, visto che le vere conseguenze della crisi ancora non le abbiamo toccate con mano. La crisi di liquidità e la mancata concessione di credito alle piccole e medie imprese da parte delle banche, con l'aggravio di una domanda aggregata che stenta a risollevarsi, produrranno come conseguenza la chiusura di molte attività imprenditoriali e l'inevitabile aumento delle persone disoccupate. I dati presentano in particolar modo un aumento della disoccupazione al Sud di circa un 12 per cento Il ministro Tremonti ha annunciato nei giorni scorsi la prossima attuazione di alcune misure a sostegno del Mezzogiorno, tra cui la previsione di una fiscalità di sviluppo, oltre alla predisposizione di una banca del Sud che possa reimpiegare i depositi accolti nelle aree sottoutilizzate. Il tema della fiscalità di vantaggio (di questo il ministro Tremonti è assolutamente consapevole, visto che ha corretto il tiro abbandonando l'idea della fiscalità di vantaggio e parlando piuttosto della defiscalizzazione dei depositi bancari al Sud,

sarà sicuramente oggetto del boicottaggio imposto dalle immancabili perplessità della coalizione di Governo. Inoltre, il provvedimento sullo scudo fiscale, definitivamente approvato alla Camera, contiene una serie di elementi fuorvianti e di indubbio cattivo gusto, ai limiti della decenza, come l'introduzione della protezione per chi usufruisce della misura della tutela contro reati gravissimi come il falso in bilancio.

e i principi etici, non si è accorto verosimilmente che tutto ciò che fino ad oggi ha detto si scontra in maniera violenta ed evidente con i principi «etici» contenuti nel cosiddetto scudo fiscale. Non si spiega altrimenti, in questo contesto, il concepimento di una norma salva evasori, che all'inizio era stata disconosciuta dal Governo,

un valore inconcepibile in un periodo ad inflazione quasi zero come quello attuale. anche il fallimento dei Tremonti *bond* sia testimonianza della circostanza che le misure predisposte dal Governo evidenziano più la voglia di una propaganda, di andare sui giornali, che l'idea concreta di produrre effetti positivi. È un modo di tirare a campare, di sperare che la crisi si risolva da sola e che, una volta risoltasi da sola senza conflitti sociali e senza perdita di consensi nei sondaggi da parte del Governo, si possa tornare a ragionare sulle questioni. Tuttavia, tutto questo tempo sarà tempo perso rispetto a questioni centrali che, se affrontate oggi, renderanno competitivo il nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei; se non affrontate, così come sta avvenendo, allontaneranno l'Italia dalla competizione con Paesi come la Germania e la Francia che, grazie alle riforme strutturali che in passato hanno fatto, alla loro dotazione infrastrutturale

che da sempre sosteniamo debbano essere oggetto di misure da parte del Governo: intanto, per quanto riguarda le politiche per la famiglia, e in particolar modo per il quoziente familiare, che è la migliore riforma che vi possa essere del sistema del welfare;

fine il conto lo paga il cittadino contribuente, o attraverso la tassazione occulta o attraverso l'inefficienza complessiva del sistema dello Stato, e in questo contesto il conto lo pagano i soggetti più deboli, cioè le famiglie italiane monoreddito e le persone disoccupate, soprattutto quelle del Mezzogiorno d'Italia.

chiunque viva e conosca la realtà di tutti i giorni non ha bisogno di dare la giusta interpretazione ai dati, alle cifre, ai saldi contenuti nella Nota di aggiornamento al DPEF per comprendere che la crisi sta tuttora colpendo duramente il nostro Paese. Questa verità non è un'invenzione di un'opposizione anti italiana o di una piazza faziosa, né è un'invenzione dell'opposizione aver sostenuto sin dai primi provvedimenti del 2008 - e ripetuto oggi sino alla paranoia che è stato irresponsabile prima e lo è ancor di più ora sottovalutare di questa crisi gli effetti negativi sull'occupazione, sui redditi bassi, sul risparmio delle famiglie frutto di sacrifici e non di speculazioni, sulle imprese in lotta per la sopravvivenza, costrette prima a licenziare e poi a chiudere. È una realtà i cui dati esatti nella loro intensità e durata nel tempo ancora sfuggono a molti, così come di certo sfuggono al Governo che, in un'ennesima occasione perduta, si ostina a non prevedere al momento alcun ulteriore intervento, né sulle politiche di bilancio, né sulle risorse impegnate e neanche sui saldi, dopo il confuso e contraddittorio intervento avviato con il decreto-legge anticrisi dell'estate scorsa. Oggi il Governo, a nostro giudizio per insipienza e mancanza di coraggio, si limita a prevedere solo un leggero ritocco per il 2010, anno che dovrebbe prevedere, secondo le sue previsioni, sistematicamente sbagliate, un saldo in leggero miglioramento. Ci è stato ripetuto che quella varata dal Consiglio dei ministri dovrebbe essere una finanziaria superleggera senza manovra, che mobilita nel triennio poco più di 3 miliardi tre articoli e relative tabelle, che si limitano ad integrare con il 2012 la manovra biennale varata nell'estate del 2008. zero tagli e zero tasse ha dichiarato il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti. Noi aggiungiamo: zero idee, zero proposte, zero azioni risolutive. Non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo accettare che si cerchi di far credere agli italiani quanto si vuole ostinatamente far apparire da una lettura distorta dei dati contenuti in questa Nota aggravati da un ottimismo mediatico e da una pratica economica illusionista, diventata ormai abile nello spostare sempre le stesse risorse. Quello che per la stragrande maggioranza dei Paesi passerà alla storia come la crisi più grave e devastante dal dopoguerra ad oggi, per Berlusconi e Tremonti è stata invece la crisi più rapida, più veloce, più indolore, un vero miracolo italiano.

(sue testuali dichiarazioni): «Negli ultimi due o tre mesi si sono ripetuti segnali non negativi per l'economia mondiale e per quella italiana». Poi, ancora, nella Nota di aggiornamento al Documento mentre le imprese chiudono i battenti e le cronache ci parlano di operai disperati sopra i tetti e di pensionati che rubano ai supermercati perché non hanno soldi per arrivare a fine mese, il Governo dichiara: «In estate il clima economico è nettamente migliorato».

considerato che l'occupazione reagisce sempre con ritardo all'andamento dell'economia e visto che molti lavoratori hanno già esaurito la durata massima dei trattamenti di cassa integrazione. Non possiamo farlo per le imprese, per quei 4.320.000 imprenditori alla guida di aziende con meno di 20 addetti che occupano circa 10 milioni di lavoratori, il 52 per cento del totale degli occupati. piccole e medie imprese che chiedono meno burocrazia, meno tasse, più credito e vogliono che i banchieri facciano semplicemente il loro vero mestiere e che, invece di trincerarsi dietro l'alibi dei numeri per poi dire un no, guardino i loro progetti, la loro volontà di intrapresa, la loro credibilità;

e di tempo se ne è perso già abbastanza! Non possiamo farlo per il Mezzogiorno dove, dopo gli annunci lanciati dal Governo, non si è fatto nulla, o meglio si sono spostate risorse dal Sud verso il Nord come sta dimostrando la tragicomica ripartizione delle risorse economiche dei fondi FAS. Il rapporto SVIMEZ, presentato il 16 luglio scorso, nel confermare che il divario tra le due Italie non solo non è stato eliminato ma in un certo modo si è aggravato, ha avuto se non altro la capacità di svegliare le forze politiche del centro-destra sulla questione meridionale, anche se le reazioni cui abbiamo assistito sono state quanto meno improvvisate. Si è parlato di ritorno delle gabbie salariali, di banca del Sud, di partito del Sud, di piano Marshall per il Sud e chi più ne ha più ne metta. Un fatto è certo: di fronte alla recessione tutti i Governi hanno modificato i loro programmi e l'Europa sa bene che i piani anticrisi in qualche modo hanno dei costi e vanno finanziati. Nel nostro Paese la finanza creativa è riuscita a far pagare gli interventi anticrisi alle aree più deboli e ha puntato per far cassa nell'immediato su operazioni vergognose, come il rientro anonimo ed agevolato di capitali accumulati illegalmente illegalmente all'estero, lasciando intatta l'imposizione sui redditi da lavoro e non toccando la leva fiscale. Gran parte dei Paesi europei ha varato manovre anticrisi basate su stimoli fiscali: lo hanno fatto la Spagna, la Francia e la Germania.

difficile spiegarlo ad un modesto lavoratore dipendente, che contribuisce con oltre il 40 per cento con le imposte dirette, rispetto a chi percepisce redditi di capitale di decine di milioni di euro all'anno e paga le imposte con un'aliquota che può essere anche inferiore al 14 per cento.

dobbiamo fare uso di un nuovo vocabolo, di una nuova terminologia, quella cioè della esclusione sociale, quella della nuova povertà, che non è solo monetaria, ma è riferita all'esclusione di un pieno godimento nella propria vita individuale e familiare dei diritti sociali e politici. Su questa linea di indirizzo si basava la cosiddetta strategia di Lisbona 2010, che avrebbe dovuto portare tutti i Paesi europei, e l'Italia tra questi, verso una piena e completa inclusione sociale. Avrebbe dovuto, perché il 2010 ormai è arrivato e la piena e completa inclusione sociale è svanita da questo orizzonte temporale. per colpa della crisi, ma anche per una politica rinunciataria; infatti, se al posto del gioco delle tre carte con i fondi FAS o di spendere miliardi con Alitalia, SCIP 2, Ponte di Messina, o spendere e spandere chiacchiere con Robin tax e Tremonti *bond*, avesse realmente impiegato risorse per dare lavoro al Sud, alle famiglie, alle piccole imprese, oggi ci sarebbero meno disoccupati, meno malessere sociale. Signor Presidente, potremmo riassumere le ragioni del nostro voto contrario alla politica economica di questo Governo in queste poche parole: «Le due metà del mondo tremontiano, il filosofo dell'economia e il furbetto del governino, sono in guerra e divise da un astio che la pratica del potere non placa, anzi di giorno in giorno accentua. Bisogna riconciliare Giulio con Tremonti, il moralista con il manovratore di scudi fiscali, il fustigatore della mala finanza con il Ministro che piace ad evasori, truffatori e falsificatori di bilancio aziendale». Queste parole, signor Presidente, signor Vice Ministro, non sono di Antonio Di Pietro, del tribunizio Antonio Di Pietro, come è stato apostrofato in alcuni casi. Non sono parole dell'eversivo Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori. Non sono le parole di una piazza aizzata e scalmanata. Sono semplicemente le giuste, attente e serene critiche della rivista «Famiglia Cristiana».

in queste riflessioni, i sentimenti e gli umori del nostro Paese, stanno cambiando.

interconnesso, nel quale ovviamente non ci siamo estraniati e stiamo facendo un'azione assolutamente positiva e propositiva. Non è mai successo, a mia

di Stato se non coperti da importanti contributi del Fondo monetario internazionale e di altri Paesi. Sicuramente in Paesi più piccoli rispetto al nostro - penso all'Islanda, ad

se non coperta da importanti contributi internazionali, avrebbe portato a situazioni complesse, che già stanno vivendo se non addirittura tragiche.

ovviamente consapevoli che nei prossimi anni, nel prossimo decennio, vi sarà una grande sfida internazionale, in particolare dei Paesi industriali,

probabilmente per questa crisi, scoppiata improvvisamente all'inizio dell'attività di questo Governo e di questo Parlamento,

Ciò riguarda sicuramente il federalismo in tutte le sue forme, da quello fiscale, già approvato, ma dovremo parlare anche di federalismo di tipo costituzionale ed altro.

Di ciò sono sicuramente consapevoli il Governo e il Parlamento e su questo ci stiamo muovendo con delle manovre sicure e certe. È ovvio che in questa fase bisogna, come dicevo prima,

Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, non entro nel merito degli aggiustamenti al margine che la Nota di aggiornamento introduce in alcune grandezze macroeconomiche, del resto non sempre adeguatamente motivati, come segnala il nostro Servizio del bilancio. Ci interessa invece esprimere un giudizio politico sintetico. Il Documento conferma la linea per noi profondamente sbagliata adottata dal Governo - in modo elegante,

È una linea doppiamente sbagliata. È sbagliata perché non si tratta di una parentesi in un processo di crescita, ma di un profondo mutamento dentro l'economia globalizzata. Nulla sarà più come prima dal punto di vista delle opportunità dei mercati, delle ragioni di scambio e delle opportunità geopolitiche per il sistema Paese e per le nostre imprese. sbagliata, perché le conseguenze sociali, in termini di perdita di lavoro, si prolungheranno ben oltre il punto di inversione della congiuntura. Naturalmente per riempire questo vuoto di azione si possono introdurre all'opinione pubblica varie distrazioni. Si fa una polemica contro gli economisti, incapaci di prevedere l'evoluzione futura: ma se noi volessimo fare una polemica sul punto, quante cifre potremmo indicare, tra quelle date da questo Governo, dimostratesi nel tempo completamente inaffidabili? Oppure ci si addentra in una sorta di

Vegas, non vanno giudicate in base all'estetica, ma in base alla capacità di approntare in modo efficace la necessità di riorganizzare la priorità della spesa, le politiche di sviluppo e la tenuta dei conti. Non c'è nulla di più leggero del nulla, ma il nulla è, appunto, la rinuncia all'azione virtuosa e coraggiosa.

vice ministro Vegas, intervenire in un momento di crisi, ma voi avete fatto questa promessa irresponsabile. La pressione fiscale è più elevata di quella lasciata in eredità dal nostro Governo, con una differenza: avete aggravato le diseguaglianze. Infatti, i redditi più bassi non hanno avuto alcun alleggerimento, mentre quelli più alti parecchi, a partire dal regalo dello scudo fiscale, in base al quale il contribuente disonesto paga meno di un quinto di quello che paga un risparmiatore che ha tenuto i soldi in banca, al servizio del Paese, o di un lavoratore che, dopo una vita di lavoro dipendente, sulla sua liquidazione continua pagare il 27 luogo, la spesa pubblica corrente continua a crescere in assoluto ed in percentuale rispetto al PIL (più 2,4 punti), pur pur avendo potuto usufruire di un forte calo delle spese di servizio del debito. Si tratta pertanto della seconda promessa mancata, poiché non c'è alcuna azione di riqualificazione della spesa né di un suo orientamento verso l'investimento. terzo luogo, inevitabilmente si deteriora gravemente l'equilibrio di bilancio, e il rapporto debito-PIL tocca il vertice del 115,1 per cento, con un incremento di quasi 10 punti in un anno, anno, nonostante si sia potuto usufruire di un forte risparmio nel servizio del debito (oltre 6 miliardi di euro). Ma fino a quando potremo contare su un costo del denaro così favorevole? il debito cresce non per finanziare attive politiche di sviluppo capaci di generare crescita più elevata, ma per automatismi che il Governo non riesce a contrastare.

che il Governo ha fatto nel dibattito estivo. Dov'è il piano per il Mezzogiorno? Dove sono le politiche attive per il lavoro e gli interventi promessi per la contrattazione di secondo livello,

Il Governo sceglie invece di vivere alla giornata affermando che comunque l'economia incomincia a muoversi. Ce ne rallegriamo e speriamo di tutto cuore che questi timidi segnali si rafforzino. Resta però il fatto che, nei primi sei mesi dell'anno, l'Italia ha fatto segnare il risultato peggiore di tutto l'Occidente in termini di calo del PIL

tutte le previsioni indicano che è un'emorragia che continuerà. Resta ancora il fatto che la cassa integrazione è cresciuta di oltre l'800 per cento in un anno. Sarà un bene se ci muoveremo più velocemente, ma dobbiamo risalire un fosso molto più profondo. questa la profonda contraddizione del Governo: il ministro Tremonti, nella sua versione letteraria, quando scrive, o nella solennità dei vertici internazionali, richiama giustamente il fatto che stiamo vivendo un passaggio d'epoca e che bisogna correggere gli eccessi del mercatismo (di cui naturalmente nel mondo è stata alfiere la destra, non certo la sinistra) sottolinea che c'è una svolta strutturale da affrontare. Ma, quando fa il Ministro, dimentica tutto ciò e rinuncia ad impostare una politica economica coraggiosa; spera che aspettare sia sufficiente. Io apprezzo sinceramente le parole che il Ministro ha pronunciato ieri sulla necessità di essere prudenti nel valutare l'entità e la stabilità della ripresa e sono consapevole della difficoltà del suo lavoro. Bisognerebbe però che quando siamo noi a ricordare che occorre essere prudenti non ricevessimo gli insulti di un Presidente del Consiglio a corto di argomenti. Vorrei poi sottolineare che esiste una certa differenza tra la virtù della prudenza ed il vizio dell'ignavia. Il nostro Paese era affetto da una sindrome da bassa crescita prima della crisi e non c'è nessun automatismo che possa riportarci a crescere più velocemente degli altri. Anzi, il quadro competitivo è molto più complicato. Qui il Governo rinuncia incomprensibilmente a misurarsi con l'attuazione di riforme coraggiose, ad incoraggiare e sostenere i nostri imprenditori, a riorientare il sistema produttivo. Faccio un solo esempio: nei giorni scorsi il Governo francese di centrodestra ha finanziato un piano, per 4 miliardi di euro, per mettere in circolazione 2 milioni di veicoli elettrici al 2020,

Ma lei non parla soltanto per sé, parla anche per chi la vuole ascoltare, e coloro che non vogliono ascoltarla dovrebbero smettere di fare questo chiasso! sto pensando ai molti radioascoltatori che ci sentono, con maggiore curiosità e attenzione forse di chi è pagato per stare qui. mentre il Governo francese fa questo, noi ci attardiamo a pietire in sede europea, senza alcun successo, modifiche peggiorative degli accordi sul clima, dopo che all'Aquila abbiamo detto che prenderemo impegni più rilevanti. Alla fine, in Francia vi sarà una industria automobilistica ammodernata e noi staremo a piangere. È la differenza tra un Governo che governa e un Governo che aspetta che passi la nottata. Eppure è un Governo di centrodestra! Ma per far tornare la luce occorre unire le migliori energie, occorre aiutare gli innovatori, occorre sul serio essere riformatori

Signor Presidente, signor vice ministro Vegas, onorevoli colleghi, inizio il mio intervento dichiarando da subito che il Gruppo del PdL del Senato darà il proprio pieno sostegno al Governo, votando a favore della proposta di risoluzione a prima firma Gasparri sulla Nota di aggiornamento al DPEF: pieno sostegno al Governo e all'impegno che in questi mesi è stato profuso dall'Esecutivo, in una crisi finanziaria ed economica di grandi dimensioni come quella che stiamo vivendo, e che secondo molti indicatori va verso una graduale e gracile ripresa. Tutte le regole economiche, finanziarie e di bilancio degli anni passati in questi mesi sono saltate, portando ad una crisi di dimensioni planetarie. I risultati del Governo Berlusconi sono sotto gli occhi di tutti, e la strada intrapresa nei mesi scorsi per la soluzione della crisi, con interventi a favore dell'impresa privata e degli ammortizzatori sociali, è stata giusta e lungimirante. Il Governo ha cercato di garantire le condizioni di stabilità per la finanza pubblica e il contenimento della spesa pubblica; ha agito al fine di salvaguardare il sistema creditizio ed il risparmio delle famiglie, sostenere i redditi e i consumi, di estendere e rifinanziare gli ammortizzatori sociali, di potenziare e accelerare gli investimenti pubblici, di incentivare gli investimenti privati.

Gli elementi emersi dalla discussione di questo documento ci danno conferma del miglioramento nell'ultima parte dell'anno in corso. Certo, la pesante situazione relativa all'interscambio relativa all'interscambio con l'estero rappresenta l'elemento centrale per comprendere la determinante più volatile, affianco agli investimenti ed all'occupazione, che causa la flessione del PIL. Chiara è anche la situazione internazionale. La crisi è essenzialmente connessa ad un pesante squilibrio delle reali partite correnti e al deficit degli USA, sterilizzati per anni da una finanza creativa senza controllo. D'altronde tutto ciò ci è molto chiaro. Se questa è, in estrema sintesi, la diagnosi, molta meno chiarezza sulle prognosi vedo da taluni proporre, anche in questa Aula, in contrapposizione con l'azione del Governo. Il riequilibrio dell'economia reale sarà ovviamente graduale, come è inevitabile che sia. Lo conferma anche l'ultimo rapporto del Fondo monetario, quando sottolinea che la recessione mostra segni di aver toccato il fondo, ma aggiunge anche che la ripresa rimarrà lenta e fragile. Pensare dunque che questa maggioranza sia responsabile, da un lato, di un calo della domanda estera è evidentemente una polemica strumentale. E, sicuramente, dall'altro lato, non possiamo uscire dalla crisi con una ulteriore e semplice espansione del deficit pubblico. Reclamare maggiore spesa pubblica significa guardare a questa crisi con impostazioni tradizionali, con lo sguardo rivolto all'indietro, a regole saltate con la crisi di questi anni. allora notiamo la singolare contraddizione delle critiche al nostro operato: ci si accusa di non adottare misure anticicliche di politica economica, nonostante proprio la spesa corrente del quadro programmatico torni a crescere nelle sue rigide determinanti nel 2010 e nel 2011. ci accusate che la nostra politica di bilancio sarebbe prociclica e, dall'altro, ci additate la situazione dei conti pubblici che peggiora per effetto del calo della crescita. La realtà è che il Governo sta usando la necessaria cautela e prudenza. Imboccheremo la fase di miglioramento senza deteriorare la finanza pubblica oltre il limite di sopportazione dato dalla credibilità del Paese sui mercati finanziari internazionali. Troppo spesso, anche in questa Aula, si tende a ragionare con il metro del passato, in anni in cui era ritenuta sostenibile qualsiasi espansione del debito pubblico e confidando soprattutto sulla certezza che il debito era sottoscritto dai risparmiatori privati interni. Questo non è più così: ormai da molti anni, circa la metà del nostro debito pubblico è collocato all'estero. A questi mercati dobbiamo rendere conto ogni giorno, ogni ora che passa. Misure espansive unilaterali rischierebbero oltretutto di allargare il famoso «effetto di spiazzamento» del settore privato. Non appena il miglioramento congiunturale ce lo permetterà, dovremo riprendere la nostra strada maestra, la riduzione del livello della pressione fiscale, e dovremo agire gradualmente sulla nostra spesa pubblica. Quando il fisco è già tanto pesante, infatti, piuttosto che creare deficit aggiuntivo nel breve termine è meglio pensare a tagliare le tasse in maniera incisiva. Le risorse provenienti anche dallo scudo fiscale ci consentiranno di finanziare ulteriori interventi anche più strutturali. Dopo gli interventi congiunturali attuati con i decreti anticrisi e il rifinanziamento della CIG, guarderemo al prossimo futuro e dovremo accelerare la ripresa che si profila già all'orizzonte. Con responsabilità dobbiamo allora confrontarci con i ritardi strutturali storici del Paese, quelli che vanno ben oltre questa recessione e che dipendono dal basso potenziale di crescita dell'economia. Queste sono scorie antiche di decenni di consociativismo che ci hanno ostacolato nella nostra azione per cambiare l'Italia. Occorre rilanciare la produttività e il differenziale di competitività del Paese. Per questo, dobbiamo agire con molta più forza per affrontare gli impedimenti strutturali alla crescita che gravano sull'economia italiana. Dobbiamo proseguire anche nelle liberalizzazioni. Con il cosiddetto collegato energia, abbiamo segnato un importante passo in avanti; sono certo che ne seguiranno molti altri. Dobbiamo farlo con una attenzione particolare al Sud. La discussione delle mozioni sul FAS, fatta in questa Aula, ci ha ricordato, ove necessario, quanto sia difficile fare impresa nel Sud. Tornare a crescere per il Mezzogiorno è una questione nazionale. Ben venga dunque una cabina di regia che coordini i mille rivoli delle risorse aggiuntive, sia nazionali che comunitarie, ed una fiscalità di vantaggio estesa che veda prioritariamente una contropartita di tipo occupazionale da settori quali il turismo, l'agricoltura e l'industria.

Non smarriamo la rotta dei nostri ideali, non cadiamo nella trappola del pessimismo, non facciamoci deviare dalle polemiche strumentali. La crisi economica resta seria. L'Italia ce la può fare se ci concentriamo se ci concentriamo su pochi obiettivi prioritari unendo tutte le intelligenze produttive e politiche. Per tutti questi motivi, e per gli obiettivi che abbiamo di fronte, votiamo a favore della proposta di risoluzione, votiamo a favore della ripresa.

le comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, saranno rese all'Assemblea

il provvedimento è molto semplice, anche se è collegato ad una vicenda tragica che stiamo ancora vivendo sulla pelle degli aquilani e degli abruzzesi e che ha impegnato, impegna ed impegnerà l'intero Paese. Si tratta del rinvio ulteriore del termine per le elezioni amministrative in Provincia dell'Aquila all'ordinario turno del 2010.

giorno, da stabilirsi dal Ministero dell'interno, tra il 1° novembre ed il 15 dicembre di quest'anno. Il Governo ha pertanto ritenuto (proprio perché siamo in una fase ancora fortemente

infatti una serie di attività sia da parte delle istituzioni pubbliche, che da parte dei partiti politici, con l'impegno di tutte le cittadinanze, che magari in questo periodo sono occupate a risolvere i pressanti problemi quotidiani che le assillano. Voglio solo far presente, come curiosità, che nel provvedimento è previsto anche il ricorso al ballottaggio per un Comune della Provincia dell'Aquila, San Benedetto dei Marsi, perché nel turno elettorale del 2008 in quel Comune si realizzò un pareggio. In quel Comune si vota a turno unico, ma dopo un ricorso al TAR, confermato dal Consiglio di Stato, si è verificato che si è realizzato un perfetto pareggio. Il nostro Testo unico sulle sulle autonomie locali prevede in materia elettorale che in questo caso si faccia luogo a un ballottaggio. La decisione finale del Consiglio di Stato è recente ed è citata nella relazione del Governo; è stata depositata il 2 aprile 2009. Quel Comune fu inserito appunto nel turno turno novembrino e adesso scivola nel turno ordinario. Certamente la situazione è singolare perché si arriverà al ballottaggio dopo due anni dal

volevo ricordare - come dicevo all'inizio - che sull'urgenza non vi è stata alcuna problematicità, che anche la parte emendativa è stata contenuta e di questo ringrazio tutti i colleghi della Commissione. C'è stata una correzione soltanto nel titolo del disegno di legge, che forma oggetto di un emendamento

che a tutt'oggi, nonostante i lavori procedano con sollecitudine e con efficacia, risulterebbe ancora particolarmente complicato e complesso

invernale che dalle nostre parti, in particolare in questa Provincia, si presenta sempre particolarmente rigida. È quindi È quindi giusto e sensato pensare ad un accorpamento con il turno naturale del 2010, previsto per la primavera.

e invece credo che il Governo fece bene - e oggi ne abbiamo la controprova - quando scelse e decise di limitare questo rinvio esclusivamente alla Provincia dell'Aquila perché nelle altre Province, Province, come poi si è dimostrato, si è potuto tranquillamente effettuare la campagna elettorale, rinnovare a scadenza naturale gli organismi comunali e provinciali, senza senza dover fare un rinvio - come qualcuno aveva chiesto - che oggi inevitabilmente avrebbe prodotto un ulteriore rinvio. Credo invece,

accadimenti che prima ricordava, anche per una razionalizzazione del sistema e della campagna elettorale. a mio avviso non logico e non di buonsenso - lo ribadisco - magari far votare qualche Comune a novembre per poi richiamarlo alle urne a marzo per le provinciali. Un unico turno elettorale, elettorale, unitamente alle altre amministrative che nella Regione Abruzzo si terranno nelle varie Province - c'è un capoluogo di provincia, come Chieti, dove si andrà a votare, ma ci sono anche altre realtà importanti collegato a tutta la tornata elettorale della primavera prossima a livello nazionale credo sia la scelta più giusta e logica. Voglio quindi

importanti ma che, spostando in avanti l'orologio elettorale di qualche mese, permetterà anche alla Provincia dell'Aquila di ritornare ad un sistema di *governance* e di campagna elettorale normale, in tranquillità e nell'assoluta serenità. Una serenità che è quanto mai necessaria, soprattutto in quella parte dell'Abruzzo, per affrontare invece le tante difficoltà che ancora ci attanagliano e sulle quali nei prossimi mesi, e purtroppo nei prossimi anni, dovremo concentrarci principalmente. *(Applausi dal

non solo ispirata al buonsenso ma soprattutto necessaria. Necessaria perché abbiamo sempre detto che la ricostruzione del cratere sismico sarà un'opera forse molto più dura, più difficile e più sofferta della stessa emergenza. Lo dicono i numeri drammatici. Ieri, signor Presidente, 6 ottobre: sei mesi esatti sono passati dalla tragedia e i numeri che rappresentano quella realtà drammatica e devastata sono ancora molto presenti. Da quel giorno, da sei mesi, L'Aquila è stata colpita da 11.000 scosse sismiche; 31.974 persone sono tuttora assistite, 15.000 in alberghi, 9.000 in case private; 7.270 sono ancora allocate in 73 tendopoli. Sono numeri che parlano da sé e che fanno comprendere a tutta l'Assemblea che non vi sono oggettivamente condizioni umane, sociali e politiche per poter svolgere regolarmente e serenamente questo importante importante appuntamento elettorale. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo voluto cogliere anche questo momento per presentare all'attenzione dell'Aula un ordine del giorno un ordine del giorno che, sulla base della drammaticità della situazione, rivolge un appello e chiede un impegno al Governo su due aspetti che riteniamo dirimenti. Il primo aspetto riguarda l'Abruzzo, che, insieme ad altre Regioni, è stato sottoposto dal Governo nazionale all'obbligo di un piano di rientro del debito sanitario a partire dall'11 settembre 2008,

evidente nella programmazione della politica regionale e sanitaria. Per sei mesi, ed è giusto che sia stato così, si è in fondo atteso che il popolo abruzzese potesse determinare con la sua volontà la nuova Giunta regionale. Successivamente, dopo pochi mesi, il 6 marzo 2009,

al pari di altre ha un bilancio regionale assorbito per l'81,8 per cento dal fondo sanitario non può

al rispetto degli obblighi finali o intermedi di un piano di rientro del debito sanitario. È materialmente, tecnicamente, politicamente impossibile.

rivedere, rivisitare, rimodulare il piano di rientro del debito sanitario. Ciò consentirebbe, già solo con il risparmio sugli interessi del debito sanitario, un recupero

bensì un'attenzione razionale e una sensibilità necessaria rispetto a questa situazione drammatica. Proprio perché non chiediamo assistenzialismo, proponiamo al Governo di poter riattivare quel processo di aziendalizzazione ospedaliera universitaria che riguarda due strutture universitarie ospedaliere dell'Abruzzo: L'Aquila, che ha una grande storia

è un processo di aziendalizzazione ospedaliera universitaria già accolto e recepito con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2002 dal Governo Berlusconi;

che riesca a creare poli di eccellenza utili e necessari nella Regione Abruzzo e al tempo stesso riorganizzare e riqualificare la spesa sanitaria.

atteggiamento fazioso, perché quanto ho ripetuto in modo molto semplice oggi in quest'Aula è stato già espresso da

Mi permetto di aggiungere, signora Presidente e signor rappresentante del Governo, che all'Aquila si deve risolvere un problema tecnico non irrilevante per il quale rischieremo di non andare a votare nemmeno nel prossimo turno. la città dell'Aquila non esiste più e i quattro collegi provinciali che insistono sul territorio del Comune dell'Aquila, signor Sottosegretario, oggi sono vuoti, cioè non vi sono più i residenti che prima componevano quei quattro collegi. Si tratta di capire se si immagina che vengano ridisegnati i collegi del Comune dell'Aquila e dei Comuni limitrofi che fanno parte di quei quattro collegi provinciali... (*Brusìo)*.

ovviamente attraverso le procedure previste dal nostro ordinamento giuridico, oppure se pensa di arrivare al rinnovo del Consiglio provinciale ormai abbondantemente scaduto nell'attuale condizione, cioè in una condizione di vuoto pneumatico, in cui i cittadini

esercitato un diritto previsto dalla legge ordinaria e si è dimesso. Dal 1° settembre del 2008 quel Comune è pertanto commissariato. Il Comune di Capistrello, retto

A quel punto i due candidati sindaco si sono ritrovati in parità: si deve quindi procedere ad un ballottaggio tra i due in quanto,

signora Presidente e signor Sottosegretario, se esiste un problema che è stato approfondito correttamente dalla Commissione affari costituzionali, è proprio la procedura in base alla quale, prima della convocazione dei comizi elettorali, si deve procedere alla rivisitazione delle liste elettorali.

dal decreto-legge n. 39, che era tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2009. Correttamente pertanto gli emendamenti individuano una finestra più larga, ossia la possibilità di votare entro il 15 gennaio 2010, ove queste procedure fossero ovviamente concluse.

Marsi. Per quest'ultimo Comune, la sentenza del Consiglio di Stato impone che lo stesso corpo elettorale che ha votato nel 2008 torni al voto nelle successive elezioni di ballottaggio.

le regionali di marzo - data oggi non ufficializzata dal Governo con proprio provvedimento, ma immaginata nella terza domenica di marzo - il ballottaggio per la provincia dell'Aquila avverrebbe nella domenica di Pasqua ed è del tutto evidente che questo non è possibile.

della norma sul terremoto. Ci diceste, allora, di no, e puntualmente cinque mesi dopo vi siete presentati con un decreto-legge che contiene quanto vi avevamo suggerito. proprio se non si volesse ragionare, ricordo ai colleghi che non vi è alcuna storia politica e tradizione in questo Paese che non incentivi i Comuni a tornare al voto una volta commissariati per ripristinare gli organi politici elettivi, cioè la volontà politica dei cittadini. E in questi tre Comuni, signor Presidente, ci troveremmo, nel caso in cui si andasse a votare a marzo 2010 o a giugno 2010, in una situazione paradossale: il Comune di Celano si troverebbe commissariato da 18 mesi, nel primo caso, o 20 mesi nel secondo, quello di Capistrello da 15 o 17 mesi, quello di San Benedetto dei Marsi da 16 o18 mesi, in una condizione economica e finanziaria disastrosa. *(Applausi

mentre lo svolgimento delle elezioni europee in provincia dell'Aquila ha dimostrato, con un fortissimo dato di astensionismo - molto più forte di quello della media nazionale -,

potrebbero essere svolte per tutte le amministrative in tutto il turno ordinario nel Paese e quindi non solo e non solo e soltanto per il caso aquilano; cioè L'Aquila ritornerebbe ad una gestione ordinaria. Sono d'accordo con il collega Lusi quando nota l'anomalia di alcune gestioni commissariali che inevitabilmente si sono protratte più a lungo del dovuto, ma d'altronde l'anomalia sta in tutta la la situazione aquilana. Mi riferisco anche a quella delle amministrazioni; basti pensare che il mandato dell'attuale

con cui intende posticipare il termine della finestra, dimostra che la difficoltà ed il disagio di arrivare ad elezioni subito, anche

maggiore rispetto a quello di dover aspettare, anche per i cittadini di Celano, San Benedetto dei Marsi e degli altri Comuni che, riconosco, si trovano in una situazione anomala, non più di tre di tre o quattro mesi per arrivare ad elezioni ordinarie ed essere riportati in un turno amministrativo nazionale insieme a tutti gli altri Comuni d'Italia.

Lusi sui collegi provinciali, voglio dire che è chiaro che la situazione che lui ha fotografato ad oggi non sarà quella che si troverà tra qualche mese, quando si svolgeranno le elezioni amministrative. Riteniamo, in del Governo e della Protezione civile, che per adesso è stato in larga parte rispettato, che la maggior parte di quelle popolazioni in primavera sarà rientrata nel territorio del Comune dell'Aquila,

Quelle condizioni non garantivano le tempestività e la regolarità del complesso procedimento elettorale e rendevano particolarmente difficoltosa la scelta delle candidature ad opera delle forze politiche

in sede di conversione del decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo aveva accolto un ordine del giorno che, evidenziando le difficoltà logistiche ed organizzative, lo impegnava a valutare l'opportunità di rinviare le elezioni amministrative relative alla alla Provincia dell'Aquila, accorpandole con il turno elettorale amministrativo generale ed ordinario previsto per la primavera del 2010. In questo senso vogliamo e dobbiamo inserire in quel turno elettorale tutte le amministrazioni che rientrano nell'ordinarietà degli scioglimenti e dei commissariamenti

apre una nuova finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

della Santissima Annunziata di Chieti, altro ospedale universitario, è evidente che sul secondo capoverso il parere non può che essere contrario e quindi inviterei

in quanto modifica la normativa generale sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, laddove l'oggetto del decreto-legge è circoscritto a disposizioni di rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella Provincia dell'Aquila.

Signora Presidente, l'emendamento 1.0.1 si proponeva di recuperare una situazione che definire assurda è veramente poco. La vicenda è collegata al decreto di scioglimento del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

il prefetto ha revocato i tre commissari, previsti ai sensi della legge sullo scioglimento dei Consigli comunali, ed ha inviato un commissario unico. La vittoria della popolazione viene quindi ulteriormente mortificata da un provvedimento di commissariamento che permane.

con questa data, i senatori Lusi e Legnini ritengono di aver superato l'obiezione fondamentale e cioè che oggi non siamo nelle condizioni, considerando i termini per la conversione in legge del decreto-legge, di apprestare tutte le operazioni per votare entro la data originaria della prima proroga.

una contraddizione. Apprezzo e condivido anche le altre osservazioni del senatore Lusi: certamente, prima si va a votare, meglio è. Ma a questo punto, credo che la scelta più logica sia far ricadere tutti questi comuni,

per farli votare, di prolungare al 15 gennaio 2010 il turno straordinario previsto dal decreto-legge Abruzzo, che apriva una finestra dal 1° novembre al 15 dicembre. a nostro parere, allo spirito del decreto-legge in conversione, che prevede il rinvio delle elezioni amministrative a primavera, proprio perché non ci sono le condizioni per votare prima. non è sostenuto da una motivazione che dia conto di esigenze particolari per far votare anticipatamente questi comuni. Esso è contrastante, inoltre, con l'ordine del giorno con il quale il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di rinviare le elezioni.

Inoltre, San Benedetto dei Marsi è specificamente indicato nella relazione illustrativa del decreto-legge come uno dei comuni per i quali sussiste l'esigenza del rinvio delle elezioni.

l'emendamento serve a riportare giustizia, laddove giustizia non è stata fatta. Il caso è semplicissimo: si tratta di un Comune sciolto per infiltrazione camorristica; segue il ricorso al TAR, il quale respinge il ricorso. Successivamente viene riproposto ricorso al Consiglio di Stato, il quale accoglie le ragioni dell'amministrazione comunale e quindi la reintegra, cancellando quell'ingiusto provvedimento di scioglimento per camorra. Nel frattempo, però, l'amministrazione ha compiuto il suo periodo naturale di consiliatura, per cui non viene reintegrata ma al suo posto viene insediato un commissario ordinario. La città, privata dell'esercizio democratico di essere amministrata da cittadini eletti da essa, è da ben due anni e mezzo con un commissario, che non ha né titolo né legittimazione. L'emendamento proposto serviva a porre rimedio a questa situazione; si arriverebbe infatti all'assurdo che vota il comune sciolto per camorra, ma non vota il comune sciolto per camorra ma il cui provvedimento ingiusto è stato annullato. È una sorta di disparità di trattamento e questo emendamento serviva a riportare in parte giustizia giustizia in questa vicenda, ma soprattutto a restituire ai cittadini di San Cipriano il diritto di scegliersi liberamente i propri rappresentanti. Mi permetto quindi di dissentire rispettosamente in ordine alla improponibilità in quanto le ragioni che sostengono quell'emendamento sono più che giuste e servono a ripristinare una situazione di legittimità.

a norma dell'articolo 97, comma 3, cari colleghi, come voi sapete, il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

circostanza che il gioco democratico di questa tornata elettorale verrebbe alterato dalla dispersione del corpo elettorale, soprattutto quello allocato sulla costa abruzzese e fuori dal Comune dell'Aquila, e in una certa tensione sociale e polemica che si ravvisa si ravvisa nel territorio, per ovvie ragioni dovute all'emergenza. Esso si rende necessario anche per non intralciare il lavoro di molte figure istituzionali in questo momento impegnate nella gestione dell'emergenza. Credo che

effetti estremamente positivi per il territorio e la nostra comunità, non possa e non debba essere intaccato in questo momento da un conflitto sociale e politico che indebolirebbe anche la capacità di far diventare tali risultati ancor più importanti. Mi preme sottolineare, per quanto riguarda la classe politica del territorio della Provincia dell'Aquila, che noi del centrodestra, pur avendo oggi

superato ogni ipotesi di opportunismo politico per interessarci invece dei problemi della nostra comunità e del nostro territorio. Per questo motivo dichiaro il voto favorevole sua soddisfazione nella condivisione totale di questa scelta.

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per richiamare l'attenzione dell'Aula su un'emergenza ambientale e di salute senza precedenti che la città di Crotone sta vivendo. Il 25 settembre 2008 il tribunale di Crotone ha disposto il sequestro di 18 aree ubicate nei Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro, sulle quali, a partire dal 1999, sono state realizzate opere pubbliche con materiali considerati altamente pericolosi; 350.000 tonnellate di scorie tossiche, tra cui arsenico, zinco, piombo, indio e mercurio, sono il campionario di veleni alla base del sequestro preventivo di queste opere, tra le quali ci sono anche due scuole medie, una scuola elementare e un liceo. Questo materiale nocivo proviene dall'ex sito Pertusola Sud che, in quasi settant'anni di attività, ha prodotto 90.000 tonnellate di ferrite di zinco e di altri materiali di risulta, con relativa devastazione degli ecosistemi vicini al sito industriale; ne sono interessate falde acquifere, il mare, i terreni e i promontori collinari vicini all'ex sito. Nel corso degli anni, oltre alla mancanza realizzazione della bonifica dell'ex area industriale della città di Crotone, vi è stato anche un mancato controllo per quanto riguarda le scorie provenienti dal sito industriale Pertusola Sud. Naturalmente, come sempre, sono state presentate numerose interrogazioni, è stata avviata in Commissione sanità un'indagine conoscitiva sugli eventuali rischi per la salute connessi all'utilizzo di sostanze tossiche per la costruzione di edifici pubblici, ma non si è arrivati ad alcuna conclusione reale. È dovuta intervenire di nuovo la procura che ha diramato, il 24 settembre scorso, i risultati di alcune indagini dei test clinici ematologici, sulle urine e sui capelli fatti su 290 ragazzi delle scuole, in cui si evince che c'è una concentrazione anomala di sostanze tossiche

*(PD)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, ancora una volta, sulla grave crisi industriale che investe lo stabilimento FIAT di Pomigliano Ieri sono state annunciate altre due settimane di cassa integrazione, e ciò è estremamente pericoloso, perché restano solo tre settimane, delle 52 complessive, di cassa integrazione guadagni, dopodiché si passa alla cassa integrazione a zero ore e, come previsto dalla legge, l'azienda dovrà dichiarare se esistano o meno esuberi strutturali. Quindi, è in pericolo il lavoro e il destino di 5.000 persone, e almeno 2.000 nell'indotto. La FIAT ripete l'appello all'Unione europea per creare al più presto una copertura adeguata di ammortizzatori sociali e chiede al Governo nuovi incentivi, anche se - devo sottolinearlo - il primo provvedimento sugli ecoincentivi non è servito a Pomigliano. La FIAT continua a non spiegare quale sarà il futuro produttivo - se ve ne sarà uno - per questo stabilimento, che è un simbolo della industrializzazione nel Mezzogiorno, e quale la sua missione industriale.

cioè di venire in Aula a riferire sulla crisi del settore automobilistico, con particolare riferimento a queste realtà in emergenza, e di aprire un tavolo nazionale prima che veramente sia troppo tardi.

«Per cinque anni nel fondo nascosti bidoni contenenti idrocarburi, arsenico, piombo. Per i casalesi affari milionari». Ancora: «Le pesche sulla terra avvelenata dal clan. In cella il proprietario del frutteto»; «Così i casalesi fanno affari milionari»; «Prodotti locali, purtroppo il rischio zero non esiste»; «La mappa dello scempio resta nel cassetto». Di fronte alla grave situazione che si perpetua nella Regione Campania, dove ancora oggi vengono interrati rifiuti tossici e pericolosi

del ministro Maroni, di costituire subito una *task force* a livello governativo per i provvedimenti del caso, anche nei confronti delle amministrazioni che non fossero all'altezza dei loro compiti.

vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea il grave problema della scuola italiana. Un problema che ha interessato l'intero Paese, la mia Regione, il Piemonte, e la mia città, Novara,

201 posti per docenti e 85 per operatori scolastici e personale amministrativo. Ciò, nonostante l'aumento degli iscritti e anche di ragazzi disabili. I precari segnalano tagli sulle ore di italiano e di informatica. Le graduatorie sono inique. Non esiste più la qualità didattica. Chiedo ai ministri Gelmini e Tremonti - quest'ultimo il vero artefice della riforma - di ripristinare la situazione qualitativa, che poi è numerica. scoperte 140 cattedre nella mia Provincia, tutte cattedre di sostegno. I genitori dei ragazzi disabili chiedono interventi urgenti. Tutto ciò crea un grave disagio sociale.

«A distanza di diciotto anni da quella scelta che ha segnato la mia vita e che non rinnego, dico basta. Ritorno in Sicilia, visto che sono una ex testimone, ritorno a casa mia, dove nessuno può cacciarmi, ritorno alla mia identità che nessuno ha diritto di cancellare. Ritorno tra i ragazzi per rivendicare il diritto alla Vita. Non torno per morire ma per lottare». Signora Presidente, è quanto scrive Piera Aiello, cognata di Rita Atria, la giovane testimone di giustizia suicidatasi dopo la strage mafiosa di Via d'Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino e i giovani poliziotti della sua scorta. Piera Aiello da testimone di giustizia aveva accettato di entrare nel sistema di protezione cambiando le proprie generalità e avviando, grazie al sostegno economico previsto dal programma, un'attività commerciale in località segreta. Questo programma è stato incautamente svelato da un componente delle forze dell'ordine. Ora, Piera Aiello è senza tutela nella sua città, a Partanna, in provincia di Trapani. Signora Presidente, la mafia ha memoria lunga e non dimentica, e ciò che accade a Piera Aiello è gravissimo. È una vittoria della cultura omertosa. Chiedo, quindi, al Ministro dell'interno di attivarsi per la sicurezza e la tutela di questa significativa ed importante testimone di giustizia. La stessa cosa chiedo per l'eurodeputato del PD ed ex sindaco di Gela Rosario Crocetta. Un piano criminale, che prevedeva l'eliminazione sua e della sua scorta, è stato sventato dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Crocetta in Belgio, a Bruxelles, non ha tutela, che invece gli viene garantita in Francia, a Strasburgo. Invito, pertanto, il Ministro dell'interno ad adoperarsi ancor di più per poter far svolgere all'onorevole Crocetta il suo mandato in Europa con la giusta serenità. Nessuna superficialità, quindi, nella consapevolezza che la mafia è un'organizzazione internazionale criminale, che deve avere paura dello Stato, e non possono essere né i testimoni di giustizia, né i rappresentanti delle istituzioni a vivere con il fiato della morte per mano mafiosa sul collo.

ai quali le banche chiedono di pagare le rate sui mutui dal 6 aprile fino al 31 dicembre. Sappiamo che coloro che traggono i maggiori profitti e vantaggi delle disgrazie sono proprio i banchieri, che in questo caso di specie sembra quasi che si siano trasformati in avvoltoi e volano perfino sulle macerie per non perderle di vista. Insieme al senatore Mascitelli ho presentato numerose interrogazioni parlamentari sulla revoca dei fidi, sulla revoca delle carte di credito. Abbiamo presentato un'interpellanza urgente, la

se quel decreto-legge per l'Abruzzo contempli o no la sospensione delle rate, perché questa povera gente con un'attività economica in ripresa. È stato calcolato che coloro che hanno un capitale residuo tra gli 85.000 e i 100.000 euro e hanno avuto la casa distrutta dal terremoto dovranno mettere in conto pagamenti arretrati di interessi tra i 2.400 e i 3.000 euro

l'Assemblea del Senato a riflettere su tale tema, perché è molto grave la modalità della minaccia. Le minacce sono sempre gravi, ma questa appare circostanziata, tanto che lo stesso presidente della Repubblica, Rutelli, ha invitato la polizia a tenere alta la vigilanza, e la DIGOS ha aperto una verifica al riguardo, proprio per la natura

una nuova finestra"). La Presidenza ha preso atto di tutte le sollecitazioni e i temi proposti e si farà carico innanzitutto di sollecitare la risposta alle interrogazioni e alle interpellanze presentate sui vari temi.